ritengo necessario che oggi nell'Assemblea del Senato ci si fermi, anche solo per pochi minuti, a considerare il significato politico e istituzionale della recente assoluzione in Corte d'appello di Antonio Bassolino, accusato di peculato. Nel 2016 questa stessa accusa era stata dichiarata prescritta, ma Bassolino aveva voluto impugnare l'assoluzione perché l'assoluzione perché la voleva piena e nel merito. La Corte d'appello gli ha dato ragione e ha riconosciuto la sua assoluta innocenza, assolvendolo per non aver commesso il fatto. Fin qui, una storia italiana di ordinaria giustizia, nella quale emerge però la volontà di un uomo delle istituzioni che, sicuro della sua innocenza, chiede di essere giudicato per i suoi comportamenti nel processo e non si accontenta di essere assolto da una prescrizione che non è in grado di sciogliere il dilemma tra innocenza e colpevolezza dell'imputato. non appena il quadro si allarga, l'assoluzione di Bassolino si tramuta dal caso personale e ordinario di un cittadino, sia pure importante, in un caso politico e istituzionale di portata nazionale. Negli ultimi quindici anni Bassolino è stato assolto ben 19 volte, dopo essere stato portato in giudizio altrettante 19 volte per accuse che infangavano il suo lavoro di amministratore pubblico e la sua figura di dirigente politico. La diciannovesima assoluzione di Antonio Bassolino conferma l'onestà, l'integrità e la limpidezza della condotta di una personalità pubblica che ha dedicato tutta la sua vita a Napoli e al suo Paese. Chi conosce, frequenta ed è amico di Antonio Bassolino non aveva certo bisogno di conferme giudiziarie. Bassolino è un uomo trasparente, molto diretto e limpido; la sua onestà personale e politica è evidente in ogni suo gesto, parola e decisione. La sua diciannovesima assoluzione ha anche un considerevole peso politico perché 19 imputazioni e 19 sentenze di assoluzione non possono essere il frutto di un errore isolato o del caso: sono il segno chiaro di un potere inquisitorio usato per 19 volte con una disinvoltura che, proprio per la sua serialità, non può non far pensare a un'intenzionale volontà di persecuzione politica. Se è vero che il giudice (anche quello dell'accusa) non solo deve essere giusto, ma deve anche apparire tale, dobbiamo dire che gli inquisitori di Bassolino non sono proprio apparsi giusti. Ma c'è di più. In un'intervista di due giorni fa l'allora procuratore della Repubblica di Napoli ha candidamente ammesso che «qualche errore lo abbiamo commesso»

Che giustizia c'è quando un cittadino innocente viene chiamato in giudizio 19 volte da una magistratura inquirente che poi, dopo 19 assoluzioni, ammette essa stessa che quelle imputazioni erano frutto dei propri errori? Non è questa la sede, né abbiamo il tempo necessario per trattare del cruciale rapporto tra politica e giustizia, ma vale la pena riportare altre parole dell'ex procuratore di Napoli in carica al tempo dell'incriminazione di Bassolino. Sempre nell'intervista di due giorni fa l'ex procuratore dice: «Era il 2010 e anche se il picco dell'emergenza rifiuti era superato, le strade rimanevano ingombre di sacchetti. (intendendo noi della Procura) in che modo spingere i sindaci a intervenire, a darsi da fare, e ci venne in mente di contestare l'epidemia colposa. Funzionò abbastanza bene, servì da sprone». Sono affermazioni insieme ingenue e sconcertanti. Non è questo il senso del precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché una cosa è chiara: se un procuratore intende spingere la pubblica amministrazione verso questa o quella condotta e lo fa utilizzando il suo potere discrezionale di indagine e di incriminazione, addirittura forzando con creatività una fattispecie penale vuol dire che siamo molto lontani da quella divisione dei poteri che è il cardine principale del nostro ordinamento democratico. Dobbiamo però sapere andare oltre perché, anche in circostanze così drammatiche, la giustizia italiana ha dimostrato che c'è un giudice in grado di garantire la legalità visto che, alla fine, ben 19 giudici hanno reso giustizia a Bassolino, rigettando accuse prive di fondamento. Resta la necessità che, a partire da queste vicende napoletane, il Parlamento e il Consiglio superiore della magistratura si interroghino sul funzionamento di un sistema accusatorio che, se usato senza equilibrio e senza sobrietà, può produrre danni irreparabili, può sconvolgere la vita di cittadini onesti che, nella lunga attesa della sentenza, vengono esposti a veri e propri processi di piazza, può portare al fallimento imprese incolpevoli, con conseguenze sociali molto gravi e può persino, come nel caso di Bassolino, interferire con metodi discutibili sul buon andamento del sistema politico e istituzionale del Paese. Dalle 19 assoluzioni di Antonio Bassolino possiamo trarre qualche insegnamento. È noto che le grandi crisi, come quella che il nostro Paese sta attraversando, possono impoverire le Nazioni o possono dare loro la forza di uscirne attraverso grandi processi di riforma dell'assetto dello Stato e delle istituzioni. Oggi l'Italia si trova davanti a questo bivio: tornare a crescere o rassegnarsi al declino. I 19 processi e le 19 assoluzioni di Antonio Bassolino ci dicono che, senza una profonda riforma del nostro sistema giudiziario, ancorata saldamente al principio costituzionale della divisione dei poteri, non solo non saremo in grado di risollevarci economicamente e socialmente,

Signor Presidente, colleghi, nelle ultime settimane la Sardegna si è trovata al centro di un'indagine mediatica iniziata da una trasmissione mandata in onda da un canale della televisione di Stato. In maniera subdola e scorretta sono stati rappresentati i fatti avvenuti a cavallo di Ferragosto, riguardanti l'apertura delle discoteche in Costa Smeralda. Conseguentemente a tali notizie, la procura del capoluogo con grande celerità ha ritenuto di dover aprire un'indagine verso le massime istituzioni regionali con l'accusa di epidemia colposa. Premetto che il presidente Solinas, all'inizio della stagione turistica, quando il virus in Sardegna era praticamente inesistente, aveva richiesto fortemente un certificato di negatività, al solo scopo di tutelare maggiormente gli abitanti della Sardegna e i tanti turisti che arrivavano. tuttavia, era stata oggetto di forti polemiche e di facili ironie e, come se non bastasse, impugnata dal Governo. Vale la pena ricordare che nel periodo di Ferragosto 17 Regioni su 20 hanno riaperto le discoteche per un numero di giorni superiore a quello concesso dalla giunta Solinas. La concessione in oggetto, infatti, era stata deliberata a seguito di un ordine del giorno del Consiglio regionale votato all'unanimità, che impegnava la Giunta a deliberare l'apertura delle discoteche dall'11 al 16 agosto, ma i consiglieri dell'opposizione hanno presto dimenticato il loro voto favorevole di agosto e hanno preferito strumentalizzare l'accaduto al fine di attaccare fortemente il governo Solinas con accuse infondate e mirate a creare disorientamento e malcontenti. Fa specie che in un momento delicato di pandemia mondiale, in cui viene lesa la libertà e in cui è richiesta grande responsabilità, si preferisca fomentare l'opinione pubblica, anziché rasserenarla con proposte risolutive. Mi chiedo inoltre perché le istituzioni dello Stato, che dovrebbero infondere un senso di giustizia e serenità nei cittadini, in quanto organo al di sopra delle parti, non siano intervenute con altrettanta celerità nei confronti del Governo Conte, che, impugnando la delibera del certificato di negatività di inizio estate, ha vanificato tutto il lavoro di prevenzione che aveva reso la Sardegna Covid *free*. In questo modo, si sono creati sia le condizioni che hanno permesso al virus di diffondersi con tutta la sua virulenza sia il tentativo di rappresentare la Sardegna come focolaio e untrice, anziché vittima e parte lesa. risultato? Enormi danni economici e di immagine. Questa vicenda, cari colleghi, mi porta a fare una riflessione conclusiva: cogliere il recente invito del nostro presidente Sergio Mattarella, per cui, affinché una partita difficile come questa possa essere vinta, occorre una leale collaborazione, stando insieme con grande senso di responsabilità. *(Applausi).*